L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Signora Presidente, onorevole Ministro, riteniamo che la necessità di predisporre rapidamente l'avvio dei lavori per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, opera di alto valore strategico per la nostra mobilità e per lo sviluppo dell'intera Nazione nonché per l'intero Mezzogiorno, si collega direttamente a quella di predisporre l'avvio di alcuni importanti completamenti della rete dei trasporti viari e ferroviari nel territorio della Regione siciliana. Considerato anche che in Considerato anche che in sede di esame del DPEF così come approvato dal Senato della Repubblica in data 9 luglio 2008, nel parere della 8a Commissione sull'allegato trasporti, è stata anche approvata un'osservazione riguardante l'inserimento nella legge-obiettivo del prolungamento della linea ferroviaria veloce Messina-Palermo fino a Trapani, si chiede di conoscere il piano di interventi predisposto dal Governo per la costruzione del ponte sullo Stretto Messina come opera strategica e si chiede contestualmente di conoscere gli interventi, egualmente strategici nel panorama complessivo nazionale, programmati per il completamento e l'ammodernamento della mobilità viaria, ferroviaria ed infrastrutturale in genere nella Regione siciliana e nell'intero Mezzogiorno.

sugli investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno, in Sicilia e in Calabria, il Governo Prodi è stato chiaro e leale. il ponte sullo Stretto ha detto: «Non è una priorità. Prima bisogna realizzare delle infrastrutture per rendere la Sicilia e la Calabria moderne, per superare una arretratezza insopportabile del sistema viario, ferroviario e intermodale». E ha stanziato dei soldi, facendo in modo che una cifra enorme - si parla di ben

Queste risorse, appena il Governo Berlusconi si è insediato, sono state spazzate via. Si è cioè attuato un comportamento ingiusto e illeale e, contraddizione delle contraddizioni, questi soldi non sono ritornati a finanziare il ponte sullo Stretto, ma a coprire delle leggi di spesa che riguardano gli interessi del Centro-Nord. Vogliamo sapere quali sono le scelte infrastrutturali su queste opere utili, condivise dalle comunità locali, che ancora attendono investimenti infrastrutturali da questo Governo.

del nostro Paese, che penso siamo tutti ormai assolutamente d'accordo siano alla base delle possibilità di ripresa reale del nostro Paese. Sappiamo quanto il *gap* infrastrutturale penalizzi il nostro Paese - mi corre l'obbligo di denunciare - soprattutto al Nord, quando si parla di velocità commerciale, di capacità di spostamento delle persone e delle merci per essere competitivi rispetto agli altri Paesi europei. Non voglio sembrare fuori tema

soprattutto al Sud. Vogliamo esprimere, invece, le nostre preoccupazioni rispetto al reperimento in tempi più ristretti possibile delle risorse necessarie per realizzare molte opere che riteniamo strategiche per tutta la Nazione, opere che soprattutto devono essere realizzate al Nord e che il Nord e tutto il Paese attendono ormai da troppo tempo. L'elenco è molto lungo, per brevità

o le opere di cui è prevista la realizzazione con risorse private, come l'autostrada della Cisa, la Cecina-Civitavecchia, la Brescia-Padova, la Bre-Be-Mi. Ci fa molto piacere sapere dal ministro Matteoli che tale opera si è finalmente sbloccata, ma è necessario avere tempi certi per quanto riguarda il reperimento delle risorse e la realizzazione Le nostre richieste, per le quali ascolteremo con molta attenzione le risposte del Ministro, non devono essere assolutamente intese come rivendicazione di un territorio, quello del Nord, ma come consapevolezza che il lavoro e le risorse del Nord hanno permesso fino ad oggi a questo Paese di vivere forse ben al di sopra delle proprie possibilità e che da qui in avanti la realizzazione di tali opere debba garantire la possibilità alle nostre imprese di operare e farsi valere in un mercato globalizzato e competitivo come quello attuale. [DE

il Governo Berlusconi, con il DPEF 2009-2013, ha inserito il ponte sullo Stretto di Messina tra le priorità ìnfrastrutturali del nostro Paese. praticamente affermato che il ponte sullo Stretto si farà; ma con quali soldi, ci chiediamo noi? Vorrei ricordare che durante la scorsa legislatura l'onorevole Antonio Di Pietro, in qualità di ministro delle infrastrutture, non sciolse la società Stretto di Messina spa, altrimenti lo Stato avrebbe dovuto pagare circa 500 milioni di euro di penali alle imprese, e le risorse stanziate con il decreto fiscale 2006 (circa 50 milioni di euro) per la costruzione del ponte furono destinate per il 70 per cento alla realizzazione di strade in Sicilia e per il 30 per cento alla Calabria. Successivamente, il Governo Berlusconi ha usato questi soldi per coprire il taglio dell'ICI, senza prevedere alcuna risorsa aggiuntiva per le infrastrutture nel disegno di legge finanziaria. Intanto le strade, le autostrade e le ferrovie nel Meridione continuano ad essere sempre più precarie. I treni, ad esempio, o non si trovano o non si riconoscono più, perché o vengono soppressi (come l'Eurostar Taranto-Potenza-Roma) oppure sono dotati di carrozze sempre più sporche e fatiscenti, nonostante Trenìtalia chieda continuamente esborsi alle Regioni meridionali per mantenere servizi che sono sempre al di sotto della sufficienza. E che dire della Salerno-Reggio Calabria, per la quale non si riesce ancora a garantire la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei subappalti? E ancora, della strada statale jonica, il cui completamento attende da anni di essere realizzato? Signor Ministro, vorremmo chiarezza su questi punti, perché sappiamo che per tutte queste opere il Governo non ha stanziato di suo nemmeno un euro e per il ponte sullo Stretto - che costa più di 6 miliardi di euro - servono subito

Signora Presidente, è noto che le politiche di bilancio e finanziarie del nostro Governo in materia di infrastrutture abbiano penalizzato e continuino a penalizzare il Mezzogiorno d'Italia. Il continuo ricorso all'utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate ha di fatto depredato di risorse importanti il Sud, anche rispetto ad importanti infrastrutture. La richiesta che i Gruppi di opposizione hanno fatto di un *question time* mirato sulle infrastrutture nel Mezzogiorno ha proprio questo scopo, quello cioè di chiarire almeno tre questioni centrali su cui, signor Ministro, le chiediamo una risposta chiara. La prima questione riguarda perché l'inserimento nel Documento di programmazione economico-finanziaria può voler dire tutto e niente; perché il Governo Prodi non solo ha tolto alla società Stretto di Messina, attraverso i fondi ex Fintecna, 1 miliardo e 300 milioni di euro (che poi sono stati a loro volta utilizzati dal Governo Berlusconi per il taglio dell'ICI), ma ha anche modificato la missione della società Stretto di Messina. Quindi, di fatto, se non si fanno interventi di natura diversa il ponte non si potrà fare, perché manca peraltro una parte importante della copertura economica. La seconda questione riguarda l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per il cui completamento sono necessari 2,1 miliardi 2,1 miliardi di euro. Infine, la terza questione riguarda la privatizzazione della Tirrenia e, in particolar modo, i collegamenti con le isole italiane, la Sicilia, la Sardegna e le isole minori. In atto vi è una crisi del sistema di trasporto marittimo che porta alla necessità della privatizzazione di alcuni settori della navigazione marittima statale e regionale; vi è però il principio della continuità territoriale e la necessità il diritto costituzionale ai collegamenti con le isole minori che viene negato e rispetto al quale non c'è una presa di posizione chiara e concreta da parte del Governo. Su tali tre questioni, centrali per lo sviluppo del Mezzogiorno in Italia Stretto, Salerno-Reggio Calabria, autostrade del mare e navigazione marittima), ci vuole una presa di posizione chiara e l'indicazione di tempi certi da parte del Governo, che fino ad oggi ha parlato solo sui giornali, non facendo capire nulla a nessuno.

atti del Governo che secondo noi non avevano la dovuta attenzione alle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno ed in modo particolare per le sue infrastrutture. Qualche volta abbiamo discusso anche di un utilizzo del FAS che noi riteniamo improprio, per non dire distorto, e attendevamo con fiducia che il riunione preannunciata per la giornata di domani, potesse cominciare a dare risposte pertinenti alle aspettative di un'area del Paese importante, segnata da un divario insopportabile, ma che ha affidato a questo Governo tante speranze ricoprendolo di un consenso generosissimo che noi siamo certi non verrà deluso; quindi, riteniamo questa fase transitoria e in via di superamento. Per questa ragione, attendo di sapere se le scelte preannunciate o filtrate dagli organi d'informazione corrispondano a verità e di quale consistenza esse siano. Infatti,

non solo abbiamo un materiale rotabile da Terzo mondo, ma vi è anche una mancanza di investimenti programmati assolutamente preoccupante perché inficia la possibilità, che noi riteniamo assolutamente chiara, che il ponte sullo Stretto sia lo strumento fondamentale per attivare la piattaforma logistica integrata. Ciò vuol dire che il ponte sullo Stretto è lo strumento di connessione che pretende di avere in Sicilia un sistema ferroviario ad alta capacità assolutamente funzionale e in Calabria un sistema ferroviario assolutamente omogeneo perché quest'area terminale del Paese diventi l'avamposto del continente europeo nel sistema di scambi economici con la piattaforma africana e con quella del Medio Oriente. Ebbene, abbiamo notizie per le quali le Ferrovie dello Stato nel loro contratto di programma addirittura limitano a 80 milioni di euro gli investimenti programmati in Sicilia. Inoltre, il ponte sullo Stretto, che noi consideriamo non solo un manifesto politico-programmatico del Governo ma un'opera indispensabile, pretende certezza di finanziamenti per superare tutte le che il Governo Prodi ha determinato non solo giudicandolo non prioritario ma ovviamente distogliendo da quell'opera importanti finanziamenti. Le riporto, signor Ministro, una frase ufficiale della società Stretto di Messina: «È impegno della società avere la disponibilità finanziaria necessaria a coprire l'intero l'intero fabbisogno per la realizzazione dell'opera, quindi i 6 miliardi di euro, prima dell'apertura dei cantieri. L'obiettivo è di escludere ogni rischio che una volta avviati i lavori l'opera possa rimanere incompiuta per la mancanza di risorse finanziarie». il ponte sullo Stretto, il Governo, oltre ad avere avviato le procedure sui vincoli e ad appostare una prima *tranche* di finanziamento, ha certezza di reperimento delle risorse e quindi un programma finanziario che garantisca la realizzazione del ponte in tempi certi perché tutto il sistema infrastrutturale siciliano possa

Presidente, spero di riuscire a rispondere in maniera soddisfacente alle questioni che sono state poste dagli onorevoli senatori interroganti. Lo farò cercando di dividere il mio intervento in due parti: la prima relativa alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina; la seconda relativa alle infrastrutture, in particolare ai collegamenti stradali, ferroviari e marittimi nelle zone del Mezzogiorno, che sono state richiamate, non senza far riferimento anche alla situazione delle infrastrutture sull'intero territorio nazionale, com'è stato richiesto. Innanzitutto, signora Presidente, onorevoli senatori, intendo ribadire, a nome del Governo, che la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina costituisce un punto assolutamente imprescindibile del programma di Governo.

punto programmatico fondamentale per lo sviluppo di alcune aree del Paese, per irrobustire l'intera linea infrastrutturale d'Italia e per connetterla ai principali progetti europei al riguardo. Conseguentemente a questa decisione assunta dal Governo nel suo programma (che è stato votato dalla maggioranza degli elettori), nello scorso giugno, com'è noto e com'è stato richiamato, l'Esecutivo ha confermato l'attualità del preminente interesse pubblico alla realizzazione dell'opera

che per scelte politiche completamente diverse, compiute nella precedente legislatura dal Governo Prodi, il ponte sullo Stretto di Messina era stato escluso dall'elenco delle opere prioritarie da avviare nel quinquennio 2008-2012, come riportato nell'Allegato infrastrutture al DPEF relativo a detto periodo. Conseguentemente alla decisione del Governo, confortata dal voto favorevole, con risoluzione di entrambi i rami del Parlamento, sul Documento di programmazione economico-finanziaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto alla società Stretto di Messina, che non era mai stata sciolta dal precedente Governo (qui ci sarebbero alcune riflessioni da fare, onorevoli senatori, non solo e non tanto sul costo della realizzazione delle opere pubbliche infrastrutturali necessarie al nostro Paese, ma anche sul costo che ha avuto il nostro Paese la decisione di non realizzare opere infrastrutturali, per i costi che si sono dovuti sostenere e per il *deficit* di infrastrutture che anch'esso si traduce in un costo economico gravante sull'intera comunità nazionale), un costo economico gravante sull'intera comunità nazionale), di porre in essere quanto prima tutte le condizioni per la ripresa delle attività inerenti alla realizzazione dell'opera, che evidentemente avevano subito significativi ritardi a seguito della decisione presa dal precedente Governo. Conseguentemente alla decisione assunta, relativa all'inserimento dell'opera del ponte sullo Stretto nel Documento di programmazione economico-finanziaria, il CIPE, con una recente delibera (adottata lo scorso 30 settembre), ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento. Vorrei chiarire al senatore De Toni dell'Italia dei Valori che gli oneri per indennizzi in favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo, per un importo stimato pari a circa 5 milioni di euro (non 6 milioni, com'è stato detto), saranno integralmente a carico della società concessionaria, che vi farà fronte con mezzi propri. quindi confermare l'intendimento e la volontà del Governo di procedere sulla strada della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. I relativi oneri, com'è noto, erano stati già individuati nella delibera del CIPE n. 66 del 2003 e sono stati quantificati in circa 6 miliardi di euro. Naturalmente, la semplice realizzazione di quest'opera strategica potrebbe da sola non essere sufficiente a risolvere la necessità di infrastrutture del Mezzogiorno d'Italia. A tal fine, cercherò ora di illustrarvi le iniziative assunte dal Governo in merito agli interventi previsti nel settore stradale, ferroviario e marittimo.

tuttavia assicurare che i lavori di modernizzazione saranno definitivamente ultimati entro il 2013. Il collegamento sul versante siciliano sarà invece assicurato dal potenziamento delle autostrade Messina-Catania e Catania-Palermo; inoltre, verrà meno, senatore D'Alì, un riferimento alla tratta ferroviaria Palermo-Trapani, come diremo successivamente. In particolare, per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in prossimità dello Stretto di Messina, sono già in corso di realizzazione le opere relative ai megalotti 5 e 6. Quest'ultimo megalotto termina in prossimità della città di Reggio Calabria. Lo stato di avanzamento per entrambi i lotti è già pari al 25 per cento. Inoltre, in prossimità dello Stretto e in particolare nell'ambito della città di Reggio Calabria, è prevista la realizzazione della nuova infrastruttura autostradale che svolgerà anche funzioni di tangenziale. Quest'opera avrà la lunghezza di 5 chilometri ed è inserita nell'elenco delle infrastrutture di interesse strategico, previste dalla legge obiettivo. infine, in fase di approvazione da parte del CIPE il progetto preliminare del megalotto 5 della statale 106 ionica, da Pellaio a Melito. Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, sia sul versante calabrese, sia su quello siciliano, saranno realizzati i seguenti interventi di adeguamento dell'attuale rete. Sul versante calabrese e fino alla città di Battipaglia, in provincia di Salerno, è previsto un adeguamento dell'attuale rete ferroviaria, la cui velocità commerciale oggi, purtroppo, non supera i 100-120 chilometri all'ora. Uno studio di fattibilità della società RFI (Rete ferroviaria italiana) per la realizzazione di una linea che porterà la velocità commerciale a circa 250 chilometri all'ora è stato già definitivamente predisposto.

in questo caso il CIPE ha già approvato il progetto preliminare del raddoppio, finanziato per un importo di circa 2 miliardi di euro. Nell'ambito della stessa relazione tra Messina e Palermo è in corso di completamento il raddoppio da Messina fino a Patti; è ancora a singolo binario, a sua volta, la tratta tra Patti e Castelbuono. In alternativa al progetto del completamento tra Messina e Palermo, la richiamata società RFI ha provveduto a presentare un piano di fattibilità del raddoppio della linea Catania-Palermo;

Il CIPE ha approvato uno studio di fattibilità dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea Palermo-Trapani. Il relativo progetto preliminare, sviluppato da Rete ferroviaria italiana, proprio in questi giorni è stato posto all'attenzione della struttura tecnica di missione del predetto Ministero per 1'attivazione delle procedure approvative

Poi consegnerò alla Presidenza dati esplicativi più dettagliati sulla realizzazione di tali progetti. Per quanto riguarda, senatore D'Alia, i collegamenti marittimi a cui lei ha fatto giustamente riferimento, occorre fare due considerazioni, una una delle quali investe le competenze che, come lei sa, spettano in materia alla Regione Sicilia. La questione non è strettamente o esclusivamente connessa con l'attività posta in essere dalle società del gruppo Tirrenia, né con il processo di privatizzazione della compagnia stessa ed è utile ricordare a tal fine che sono già stati stanziati 30 milioni di euro per l'istituzione di un servizio di trasporto marittimo veloce tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Entro il corrente anno verrà stipulato il contratto di servizio con il consorzio che, una volta registrato dal competente ufficio di controllo, darà la possibilità di effettuare l'impegno dei fondi, in modo da rendere operativa la metropolitana del mare nello Stretto di Messina. D'Alia, dei trasporti nelle isole minori, voglio ricordare che la questione dei finanziamenti deliberati dalla Giunta regionale siciliana, che ha competenza in materia, è all'attenzione del Governo e che esso intende fare in modo che venga assicurata la funzione propria dello Stato di garantire la continuità territoriale attraverso il servizio espletato dalle società del gruppo Tirrenia. Come lei sa, senatore D'Alia, la società che gestisce i collegamenti marittimi interni alla Sicilia è la Siremar, che assicura una griglia di collegamenti, garantendo così la mobilità dei cittadini siciliani, con tutte le isole minori

comunque prevedono opere infrastrutturali ed interventi in settori di interesse degli enti locali, che hanno preminenti interessi nel Mezzogiorno d'Italia (come le città di Catania o di Palermo), oltre che nelle altre zone del Paese, come richiesto anche dal senatore Mura.

Ringrazio, in particolare, il Ministro per l'importante considerazione che ha inserito in ordine alla centralità mediterranea dell'intera Sicilia. La Sicilia non è solamente, come a volte viene superficialmente indicato, piattaforma logistica grazie alla sua posizione geografica: essa è il cuore, culturale e storico, del Mediterraneo; ancor prima che del transito delle merci e dei traffici la Sicilia è il luogo dell'incontro, degli uomini, delle idee e delle culture dei popoli mediterranei, ed in tale veste dovrà svolgere una sua rinnovata missione nello sviluppo della civiltà mondiale nei futuri decenni. L'istituzione, nel 2010, dell'area di libero scambio del Mediterraneo (data che il nostro Governo dovrà curare non venga procrastinata) dovrà trovare preparata l'intera Nazione italiana, e la Sicilia in particolare, per il convinto impulso del Governo nazionale, soprattutto nelle strutture, tutte le strutture dedicate all'efficienza dei trasporti.

che sino adesso il Governo Berlusconi non ha stanziato un euro per alcuna opera nuova: "faremo", "diremo", un elenco di promesse e di studi di fattibilità su opere già finanziate.

fare sentire la loro voce e rappresentare con dignità, a testa alta, sui dati certi, gli interessi legittimi e legali del Mezzogiorno e, per quanto mi riguarda, della Sicilia.

Ma noi attendiamo con fiducia di trovare insieme al Governo le risorse necessarie e aspettiamo che si verifichino tutte le condizioni per realizzare infrastrutture solo potranno garantire le condizioni per una ripresa del Nord, ma potranno rappresentare un traino per la rinascita di tutto il Paese. Noi siamo pronti, come forza di Governo, a dare - come sempre - il nostro contributo in termini di idee, di progettualità. Perché non sono io, non è la Lega Nord, ma oggi (anche attraverso la trasmissione televisiva) è tutto il Paese che ci sta ascoltando e aspetta che noi si sia in grado di dare adesso ciò di cui ha bisogno.

Grazie, e non fa altro che interrompere quel processo di recupero del livello degli stanziamenti attuato nelle due precedenti manovre del Governo Prodi, che aveva portato all'aumento di spesa per investimento del 22 per cento nel 2007 Credo non si possa continuare in questo modo, signor Ministro. Il nostro Paese ha bisogno di un serio rilancio infrastrutturale, che interessi tutto il territorio nazionale, da Brescia a Palermo (io sono bresciano). Per far questo serve la certezza delle risorse, non pseudoaccordi di facciata, come quello stipulato con la BEI, che non è un accordo di finanziamento, ma è un'intesa finalizzata ad una più tempestiva valutazione dei progetti da parte della Banca. Termino qui, auspicando un futuro migliore.

ha dovuto fornirci un quadro e una rappresentazione di un piano dei trasporti e di alcune opere che conosciamo da tempo; ci consentirà tuttavia di non essere assolutamente soddisfatti della sua risposta, perché la nostra domanda aveva un fine specifico.

ha modificato l'assetto societario della Stretto di Messina S.p.a con l'uscita di Fintecna, quindi dei capitali ad essa relativi, e ha modificato la missione della società che dovrebbe portare avanti gli adempimenti per la realizzazione di questa grande infrastruttura; cosa fa il Governo attuale per riparare a questo? Non basta dire: «Invitiamo la società a mettere in atto». Serve in primo luogo un intervento legislativo che rimodifichi la missione della Stretto di Messina S.p.a e la composizione societaria. In secondo luogo,

siccome per completare quest'opera sono necessari 2,1 miliardi di euro, queste somme ci sono o non ci sono? Sono previste o no? C'è la copertura integrale? Altrimenti l'indicazione del 2013 come termine per l'ultimazione della Salerno-Reggio Calabria diventa una pia illusione o,

solo: dovete fare con la Tirrenia quello che avete fatto con Alitalia. Siccome la Tirrenia è l'Alitalia del mare ed è l'Alitalia dei poveri, cioè del Mezzogiorno, non potete pensare di realizzare una privatizzazione a costo zero, caricando i collegamenti e le tratte sociali sul privato, che non le farà mai perché sono diseconomiche. Questa è una pura follia. Dovete rivedere la politica del Governo sulla Tirrenia

che garantisce la continuità territoriale e che il vostro Governo, la Tirrenia e la Siremar intendono dismettere, anzi, hanno già dismesso dal 1° gennaio scorso. Noi siamo in questo caso in presenza di una piena violazione di diritti costituzionalmente garantiti, che non si possono far passare con una pseudoprivatizzazione, che ha il sapore della macelleria nei trasporti pubblici e che fa tornare le isole minori agli anni Cinquanta. Di questo bisogna parlare. Voi dovete assumervi responsabilità maggiori di quelle che non avete assunto qui oggi.

La migliore conferma avverrà nei fatti, quando il CIPE apposterà le somme per poter attivare immediatamente la procedura sospesa dal Governo Prodi. L'impegno politico quindi è ampiamente apprezzabile, ma il risultato che ci aspettiamo diverrà sostanziale con il ripristino del finanziamento e con l'eventuale adeguamento per garantire il fabbisogno e dare corso alle attività concrete, visto che c'è un *general contractor* che aspetta di ricevere l'ordine di inizio attività che non ha

di finanza pubblica relativo a questa partita non violerà le tante indicazioni del Parlamento che sono formalizzate in atti legislativi che prevedono il rapporto 85

tra autonomie locali e Stato centrale: noi che siamo gelosi custodi delle autonomie locali e leali sostenitori del Governo centrale pretendiamo che nella gestione di tali risorse sia mantenuta questa corrispondenza. Le dico invece francamente che non sono insoddisfatto delle sue risposte,

culturali, economiche e sociali, che vanno connesse. È per questo che vogliamo l'Alta capacità ferroviaria tra le aree di Palermo e Catania e una connessione con Messina, affinché le aree metropolitane

conversione in legge del decreto-legge n. 10 novembre 2008, n. 180 recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della rIcerca; nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.20, 1.21, 1.24, 1.25, 1.49, 1.31, 1.32, 1.66, 1.67, 1.88, 1.89, 1.90, 1.98, 1.101, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 3.0.13, 3.4, 3.0.15, 3.5 e 3.0.14. Esprime, altresì, parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 1.19, 1.95 e 1.99. Esprime parere non ostativo, alle seguenti condizioni rese, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: - che all'emendamento 1.78 siano aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per la partecipazione all'attività della Commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica"; che agli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, dopo le parole: "modalità e criteri per la costituzione" siano aggiunte le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti, osservando che l'emendamento 3.100 recepisce la condizione resa, ai sensi della medesima norma costituzionale, sul testo».

Signor Presidente, mi rivolgo al Governo:

la natura del decreto-legge è inadeguata alla natura della materia: manca il tempo per discutere qualcosa che qui è stato considerato importantissimo per la quale materia si è detto generosamente al Ministro che è stata coraggiosa. Non ci siamo. Gli emendamenti all'articolo 1, peraltro ricco di otto commi,

di partecipare ad una riforma vera del settore università. In questa maniera abbiamo previsto

la maggioranza ad esprimere le sue perplessità con molto pudore e noi opposizione ad affermare che non possiamo essere d'accordo. I nostri emendamenti servono a preparare preventivamente un'attenzione rispetto a quando avremo una riforma vera. Questo decreto non ci convince, perché se dicessimo che ci convince alla fine rischieremmo di averlo per sempre: invece deve essere *una* *tantum*, e davvero *una*, la prima e ultima volta, che si parla di università come avviene con questo decreto. senatore Rusconi

un elemento decisivo per il futuro dell'università: si tratta invece, semplicemente, di un intervento di emergenza del quale abbiamo messo in luce tutti gli aspetti negativi ed i limiti, pur riconoscendo che in alcune parti contiene elementi di positività.

in modo improprio all'interno di un decreto‑legge in materia finanziaria, una norma - questa sì - di carattere strutturale e fondativo, che apre la strada alla privatizzazione delle università.

Presidente, ad un processo di privatizzazione una delle istituzioni fondative del nostro Stato decisa soltanto dalla maggioranza dei docenti che compongono

compreso il controllo della Corte dei conti. Non si comprende allora in alcun modo la coerenza tra una scelta di privatizzazione ed il mantenimento di tutta una normativa che scusi, le chiederei, dato che sto sollevando una questione di carattere strutturale, che ci fosse la presenza di qualcuno nei banchi Bastico, stavo per interrompere il suo intervento, poi ho visto che il Sottosegretario sta discutendo con il

di rilevanza fondamentale contenuta negli emendamenti da me sottoscritti come prima firmataria volti ad abrogare integralmente l'articolo 16 della legge n.

prefigura più un soggetto pubblico che un soggetto privato. Delle due l'una: fate una scelta chiara. Noi siamo contrari ad un processo di privatizzazione dell'università anche perché - voglio ricordarlo a questo Governo - già il Governo Berlusconi per firma del ministro Moratti, così come il Governo Prodi per impegno del ministro Mussi, hanno sempre sottoscritto a livello internazionale tutti gli atti che sottolineavano come le università siano un bene di natura pubblica perché attengono attengono al diritto all'istruzione che è un diritto fondante per le persone. Questa privatizzazione, quindi, determinata esclusivamente da una scelta dei docenti a maggioranza che compongono l'università, mi sembra davvero non condivisibile.

procedure di valutazione dei concorsi: noi abbiamo proposto una soluzione con il sorteggio secco che ci sembra l'unica in grado di impedire pasticci baronali, accordi precedenti eccetera. Il sistema di passare prima attraverso le elezioni e poi di procedere al sorteggio dà scarse garanzie.

commissari e parenti candidati. Proponiamo, quindi, una soluzione per evitare che possano fare parte della commissione di concorso professori che sono parenti dei candidati.

dell'Aula: il meccanismo della legge è concepito in maniera tale che, se le fondazioni private accedono al controllo delle università, di fatto entrano in possesso del loro patrimonio,

possa esercitare un imperio proprietario sui beni immobili in possesso originario dell'università. È facile immaginare perché. Ci sono, infatti, soltanto due possibili destini di fronte a un fatto di questo tipo: secondo una prima soluzione non meravigliosa ma sopportabile

dell'altra soluzione, che temiamo non sia lontana dalla possibilità del reale, ci potrebbero essere accordi sotterranei per cui i beni immobili vengono messi in vendita a condizioni speciali a clienti speciali e a prezzi speciali.

del 2008. Non capiamo oggettivamente come possano tornare i numeri e quali siano le prospettive o, meglio, lo capiamo perfettamente e sappiamo che questo decreto, che è stato presentato dalla maggioranza come risolutivo dei problemi dell'università, in realtà è semplicemente un palliativo o un piccolo provvedimento su alcune piccole questioni. Di conseguenza, saremo obbligati a tornare a discutere del grande ed importante tema dell'università in un momento successivo.

di laurea e, in alcune situazioni specifiche, l'interesse dell'università stessa e degli studenti. Crediamo vi si debba porre rimedio e con questo emendamento chiediamo al Governo e alla maggioranza un'ulteriore riflessione in modo che si torni,

Grazie,

con i miei emendamenti all'articolo 1 cerco di mettere in evidenza i limiti e le contraddizioni di questo provvedimento, per cui non mi trovo d'accordo con la relazione entusiastica che il Ministro ha fatto oggi, soprattutto come risposta ai problemi dell'università: onestamente di risposte non ne abbiamo viste nei quattro articoli che compongono il provvedimento. Basterebbe vedere come la Commissione bilancio stamattina, dal suo punto di vista, ha chiarito che tutti gli emendamenti approvati ieri in Commissione istruzione debbano essere senza oneri aggiuntivi; i criteri, poi, sulla buona gestione delle singole università sono molto discutibili, dal momento che sono riferiti solo alle spese del personale rispetto a trasferimenti effettivi e non a trasferimenti teorici. Questo, di fatto, penalizza le università che hanno già meno e rischiano, in questo modo, di avere ancora meno. In più, l'idea del sorteggio, presentata come soluzione di tutti i problemi, ha già rivelato tutte le sue fatiche in Commissione, dal momento che si è dovuta già cambiare perché il numero in alcune discipline era insufficiente, come insufficiente è, del resto, tutto il decreto. [LIVI

ho vinto un concorso universitario nel 1966 come professore di prima fascia, come si direbbe oggi, e dal 1970 ho fatto parte di commissioni di concorso elette con tutte le possibili varianti; sono stato eletto nelle commissioni - giudichino quelli che mi conoscono - forse per la mia capacità manovriera e baronale, ma forse anche per l'immagine di onestà che avevo presso i colleghi. le dico per esperienza che non c'è marchingegno, non c'è meccanismo concorsuale che non sia possibile aprire con algoritmi grimaldello.

Meglio sarebbe stato allora mantenere il sistema esistente, eliminando la doppia idoneità che è fonte di corruzione, oppure, come viene proposto negli emendamenti da me presentati,

già stanco carro universitario. Ritengo che sarebbe stata una semplificazione apprezzata e avrebbe cercato di eliminare gli abusi. avviso, una materia così delicata come quella del reclutamento non può essere risolta con un decreto-legge che, per l'ennesima volta, cambia i meccanismi

a questa legge va demandata la riforma del reclutamento. tra i potenziali giudici per i concorsi di seconda fascia, così come è oggi; mi sembra infatti ingiusto, con l'idea che sono sottoposti a ricatto dai professori più anziani, che professori già qualificati vengano esclusi dalle commissioni giudicatrici. mediamente tali docenti sono più giovani e più a contatto con la realtà scientifica. Anche per i concorsi da ricercatori vanno reintrodotti nella commissione giudicatrice il professore associato e il ricercatore, perché,

che dovrebbe avere carattere di urgenza, una riforma complicata per costituire l'ennesimo algoritmo di composizione di una commissione. Sappiamo che gli esiti non saranno migliori dei precedenti; tanto valeva risparmiare tempo e fatica.

50 per cento delle spese per il personale cessato dal servizio nell'anno precedente per l'assunzione dei nuovi ricercatori;

per dare il senso di un'apertura, di una universalità nei confronti dei ricercatori. Pertanto, nelle briciole che questo decreto-legge consente di recuperare

Signor Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 per rivolgermi alla maggioranza di Governo. Noi abbiamo apprezzato la replica della ministro Gelmini, ma un provvedimento di questa natura non può essere affrontato né con un decreto-legge, né comunque con un dibattito strozzato. Tralasciando il fatto che questo decreto-legge non fa altro che passare una pomatina sulle ustioni di terzo grado del sistema della formazione universitaria italiana e mettere qualche pannicello caldo, ad esempio sul sistema dei concorsi, credo che sarebbe stato opportuno affrontare

Il fatto che siamo costretti ad affrontare per decreto solo piccoli aspetti di un problema enorme, cioè come riformare il sistema della ricerca e dell'università

eliminare il meccanismo, che è una forma di mediazione tra il concorso locale e quello nazionale, che viene riproposto dal Governo con il solo correttivo di un sorteggio sussidiario. Ci saremmo Ci saremmo potuti confrontare, ad esempio, sull'ipotesi di introdurre seriamente il sorteggio per evitare che le commissioni di concorso siano pilotate. Infatti, è inutile che ci prendiamo in giro: lo saranno comunque, anche dopo che approverete questo disegno di legge, e non sarà questa piccola toppa a coprire i problemi emersi intorno al mondo dell'università italiana, in tutte le parti d'Italia. Avremmo potuto proporvi un sistema generalizzato di sorteggio senza le elezioni. È chiaro, infatti, che il meccanismo che condiziona le commissioni di concorso è quello delle elezioni preventive e della composizione con il membro di facoltà necessario in sede legale di commissione di concorso. Noi abbiamo cercato, sia all'articolo 1, sia agli altri articoli del testo del decreto-legge, di offrire piccoli contributi, perché piccolo è il testo che voi ci proponete, tanto piccolo che non risolverà nessuno dei problemi dell'università italiana. Ma anche in questo contesto non vogliamo sottrarci al confronto e formuliamo le nostre proposte: ci auguriamo che vengano prese in considerazione al pari delle altre. Non ci pare

non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica».

il parere è favorevole.

Il primo impegna il Governo ad inserire nella prossima riforma del reclutamento universitario il divieto di chiamata sul medesimo settore disciplinare di parenti entro il terzo grado, compreso il coniuge e i conviventi; e i conviventi; il secondo impegna il Governo a considerare, nella ripartizione delle risorse all'università ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le particolari specificità, in termini di qualità della ricerca svolta, di singoli dipartimenti. Sono due ordini del giorno che vanno ad aggiungersi

Per contribuire a rasserenare il dibattito e venire incontro alle esigenze dell'opposizione, ritiro l'emendamento corretto), mi permetterei di insistere, perché si tratta di una norma meramente tecnica, funzionale a risolvere questioni contingenti di ricorsi

Non deve più accadere, a mio parere, ciò che è successo oggi, ossia che non si lavori secondo regole di rispetto reciproco.

quando la seduta era già in corso. Il fax è un documento ufficiale e siamo pronti a farglielo visionare. In queste condizioni credo che ci debba concedere almeno un quarto d'ora di sospensione per fare

ci sono degli emendamenti abbondantemente noti all'Aula e a ciascun senatore. Sull'emendamento in questione, se il tempo che nel frattempo impiegheremo non basterà per un'esatta comprensione, valuteremo l'ipotesi di aggiungere altri 15 minuti.

molto brevemente per ricordare che ieri l'Aula ha interrotto tre volte i suoi lavori per esigenze del Governo e della maggioranza di chiarire alcuni ho già accolto la richiesta. Ho detto che quando arriveremo all'emendamento in questione,

e si è visto dal numero degli interventi che sono stati fatti.

sia forse dovuto al fatto che si tratta di un decreto-legge, che i tempi sono stati contingentati e probabilmente anche alla circostanza che arriviamo ad una votazione come quella di stasera in tempi ristretti, che non ci permettono un sufficiente Con l'emendamento 1.5 si cerca di modificare la norma affinché alcune importantissime e storiche università del nostro Paese

di verifica del numero legale si vota per alzata di mano, non si può più chiedere il voto elettronico. Quindi, stia calma e non si preoccupi, l'opposizione da questa Presidenza è supergarantita.

Presidente, prima lei giustamente ha suggerito al relatore, che aveva espresso ad esempio su questo emendamento il parere contrario,

Le chiedo la cortesia che le riconosco ha mantenuto finora, Presidente, e la ringrazio di questo.

che può darle tutti i suggerimenti su come votare. E non si offende nessuno perché è un segnale di gentilezza.

*(PD)*. Signor Presidente, da qui ho visto che la postazione del senatore Lusi si è illuminata automaticamente.

La seduta è ripresa. Gli Uffici della Presidenza hanno proceduto al controllo. Sono stati sostituiti due terminali e in ogni caso, a fine seduta, si procederà ad un ulteriore controllo

Grazie, Presidente!

pregare i colleghi di stare al proprio posto perché, come noteranno, muovendosi fanno soltanto perdere del tempo.

Presidente, abbiamo presentato alcuni emendamenti perché riteniamo che, se è vera l'intenzione del Governo di migliorare la qualità dell'offerta formativa e della ricerca scientifica e se gli intendimenti del Governo sono reali, bisognerebbe allora ancorare ed attribuire solo all'ANVUR la competenza per la valutazione del merito e della qualità delle università. università. La ANVUR è quella Agenzia di valutazione, quella sorta di autorità indipendente costituita nel 2006 e che non ha mai potuto da allora funzionare. Tutti i processi di valutazione sono stati bloccati e quindi si è attribuito questo compito ad altre commissioni che non hanno quel requisito di indipendenza e di autonomia funzionale ad effettuare una valutazione realmente obiettiva della qualità delle università.

né nel merito, né nel metodo, per dire che si sta ponendo in essere un sistema di valutazione della qualità delle università italiane. Si sta solo buttando un po' di fumo negli occhi. L'altra questione è che c'è un'autorità indipendente che ha il compito dal 2006 di occuparsi di tutto ciò, ma che con vari provvedimenti e con vari decreti non è mai stata messa nelle condizioni di effettuare una valutazione, cioè di svolgere le funzioni per le quali è stata istituita.

alla qualità e quantità delle applicazioni scientifiche ed industriali. Esso mira cioè a premiare quelle università che sono collegate con il sistema produttivo e il riscontro di questo collegamento è dato dalla circostanza

che siamo ai pannicelli caldi con questo decreto-legge e che, tranne un po' di spolvero per dire che ci si sta occupando dell'università, non si vuole fare altro, sia perché si interviene con decreto sia perché si interviene male, senza premiare il merito e senza incentivare quelle università che già oggi

dare un potere soggettivo abnorme, oltre che enorme, ai valutatori, come se le università, che hanno la loro autonomia, dovessero soggiacere ad un giudizio di qualità sulla loro offerta formativa: e chi lo dà il giudizio di qualità?

a mia prima firma, gli emendamenti 2.5 e 2.8. Il primo introduce altri criteri, oltre a quelli prescritti, come l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche decentrate delle università. È solo una una segnalazione con la quale vogliamo chiarire che questo articolo non è sufficiente, con i suoi tre punti, *a)*, *b)* e *c)*, per definire la qualità e il merito delle università. Approfitto di questo intervento per chiedere di aggiungere la firma all'emendamento 2.6 e ringrazio la Commissione per avere votato all'unanimità

L'ordine del giorno G2.101 impegna il Governo «a mettere in atto tutte le procedure necessarie affinché i contribuenti italiani possano trasferire l'8 per mille dell'IRPEF alla ricerca pubblica». Si tratta dello stesso tema, articolato in un modo diverso. Paese; impegna il Governo a garantire l'integrità e la salvaguardia del patrimonio universitario nazionale, anche, ove necessario, mediante l'adozione di misure volte all'inalienabilità di categorie di beni di particolare rilevanza storica, artistica, paesaggistica e culturale, nonché il pieno rispetto delle tutele previste e dei vincoli apposti ai sensi della legislazione vigenteۛ». Il riferimento è sempre alla salvaguardia del patrimonio universitario, che sappiamo essere in alcuni casi particolarmente rilevante. È quindi

Questo decreto prevede di premiare senza molti criteri il merito almeno con il 7

quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona, tenendo però presente che finanziare la ricerca in un clima e in un Paese dove esistono leggi proibizioniste che, ad esempio, non consentono quella sulle cellule staminali embrionali, è un esercizio che, da una parte, tappa un buco, ma dall'altra

ripresa. Le sto chiedendo esclusivamente un chiarimento rispetto a quanto aveva detto il presidente Nania.

Presidente, colleghe e colleghi, non so se può interessare si tratta di un argomento delicatissimo - il tema del diritto allo studio, perché di questo stiamo parlando. Con l'emendamento 3.1 si vuole rendere quel lievissimo incremento, che è proprio piccolissimo,

ma credo a tanti di noi, un po' più importante di quello, pur delicato, dei concorsi e mi sembra che questo emendamento, anch'esso utile a una causa comune, possa essere accolto,

ma con un limite molto chiaro. Questi finanziamenti non sono triennali, ma sono previsti solo per il 2009.

di fatto non incrina in nessuno modo la legge n. 133 del 2008, non solo perché la Commissione bilancio si è affrettata su tutti gli emendamenti passati in Commissione a chiarire che non vi sarà alcun onere

«Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, saranno determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individuerà gli insegnamenti da attivare».

n. 509 del 1999 paghino le tasse universitarie per fare un secondo ciclo di studi o debbano accedere attraverso procedure selettive alla frequenza di un secondo ed ulteriore corso di laurea. Ci sembra un problema di correttezza e di giustizia nei confronti di questi soggetti. L'emendamento 3.0.16, signora Presidente,

una moltiplicazione delle università nata dall'esigenza, a volte fuori luogo, di moltiplicare le cattedre. Con questo emendamento proponiamo che il Governo e il Ministro dell'istruzione, dell'università

di garanzia del diritto allo studio. È un emendamento che segnala all'Esecutivo la necessità di affrontare un nodo strutturale, perché altrimenti restiamo sempre ancorati alla logica dei pannicelli caldi.

sui ricavi superiori ai 25 milioni di euro delle imprese che si occupano di idrocarburi, andando ad attaccare - diciamo noi - ma più precisamente andando a modificare la

Passiamo all'emendamento 1.5,

Dichiaro aperta la votazione.

lezione. Siccome a me l'idea può andare bene, anche perché i radicali stanno facendo lo stesso tipo di operazione per quanto riguarda la politica, mi asterrò e non parteciperò al voto, altrimenti dovrei esprimere un voto contrario.

Prego, senatore.

e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle Istituzioni individuerà gli insegnamenti da attivare.».

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1197, recante conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, in materia di diritto allo studio, valorizzazione del merito e qualità del sistema universitario e della ricerca impegna il Governo a prevedere, per gli studenti universitari fuori corso per oltre due anni accademici che non siano studenti lavoratori all'atto dell'iscrizione

potrebbe tuttavia affrontare con maggiore legittimità il problema degli studenti fuori corso - che qualche volta esagerano - se lo Stato italiano avesse preventivamente avuto la capacità di fornire agli studenti meritevoli ed anche a quelli in condizioni critiche

Un'abitazione a basso prezzo soprattutto, perché non possiamo trascurare il fatto che basta entrare in una qualsiasi facoltà per vedere che i posti letto costano da 350 euro in su. in su. In una condizione di maggiore giustizia sociale si potrebbe anche discutere della penalizzazione degli studenti fuori corso,

dobbiamo fare demagogia ad ogni costo e capisco che dobbiamo perseguire i fannulloni anche quando sono fuori corso, però questo ordine del giorno, se lo leggete con attenzione, crea due effetti contrari.

di studenti fuori corso, in molte università, pur di avere meno studenti fuori corso, non si dà più il 18 politico ma il 30 politico, per mantenersi in alcuni parametri sbagliati. L'idea di introdurre un ordine del giorno di questa natura, che non differenzia le varie posizioni soggettive,

Ci sono delle ragioni di cortesia che vanno anche oltre la lettera del Regolamento e che noi complessivamente abbiamo in questa giornata concesso all'opposizione: ci deve essere riconosciuto.

anche nella considerazione dell'orario di chiusura dei nostri lavori. Abbiamo lavorato bene ed intensamente e credo che vi sia la legittima aspettativa di arrivare al voto finale.

Signora Presidente, quello che stiamo per votare è un emendamento sul quale il Governo verosimilmente avrebbe potuto riflettere un po' di più. Noi chiediamo che il Ministro si faccia carico di predisporre, d'intesa con le Regioni e con l'ANVUR, un piano di riduzione delle università italiane tenendo conto della dislocazione regionale, della garanzia fondamentale del diritto allo studio e soprattutto dell'accorpamento di quella moltiplicazione delle cattedre che tutti noi a parole contestiamo. Tutto ciò non da domani, ma attraverso un dialogo ed un percorso che dura tre anni e tenendo conto del fatto che bisogna garantire le varie realtà territoriali. Poiché mi era parso di capire dalle dichiarazioni del ministro Gelmini che lo scopo di questo piccolo decreto è quello di andare incontro ai problemi, tentando quindi di razionalizzare, di evitare le baronie, i privilegi, le incrostazioni e quant'altro, l'idea di cominciare un percorso riformatore dell'università che punti alla riduzione

senatore Rusconi.

Quello che è stato detto prima l'ho chiesto anche come chiarimento ai due Presidenti; quello che è stato detto prima anche dal relatore, al momento... *(PD)*. Non è un problema di voce, ma di microfono, Presidente. Noi non abbiamo protestato su un fatto abbastanza inconsueto e cioè che il relatore abbia presentato

Presidente, in continuità con l'atteggiamento mantenuto, se ci viene garantito che chiudiamo i lavori questa sera e che possiamo svolgere le dichiarazioni di voto - che, tra le altre cose, come maggioranza ci impegniamo a limitare al minimo - siamo

emendamenti che riguardano un settore così importante. Credo che non accada nulla di grave se per dieci minuti sospendiamo i lavori dell'Assemblea.

infatti, che le dichiarazioni di voto non siano importanti, visto quello che ha detto il Ministro oggi, anche se purtroppo ora non è qui a sentire. Magari martedì il Ministro potrebbe essere presente.

signora Presidente, che noi avevamo acceduto alla possibilità di questo approfondimento, ma con l'impegno di andare avanti, perché è vero che il provvedimento è importante, ma se è importante, a maggior ragione, tanto vale votarlo questa sera e non fare un ostruzionismo inutile fino a martedì.

per la verità ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso, ma questo poco importa. Mi preme sottolineare, senatore Gasparri, che, ad esempio, c'è un emendamento della Commissione che credo dovreste leggere anche voi, perché altrimenti finiamo tutti sui giornali:

prendo la parola semplicemente e molto brevemente per dare un po' di trasparenza ai nostri rapporti.

Abbiamo avuto dal presidente Nania la garanzia che per alcuni emendamenti che erano stati presentati nel corso della seduta sarebbe stato dato un brevissimo tempo ai nostri Gruppi per poterli esaminare. Credo che sia assolutamente legittimo ed auspicabile che i partiti di maggioranza riducano i loro interventi di tutto il tempo necessario.

quindi il tempo materiale per confrontarci con il testo. Siamo tutti abituati a confrontarci con i testi, ma i testi di legge sono diversi, non hanno la trasparenza filologica di un testo scientifico. Quando ci troviamo di fronte ad una sostituzione di questo tipo, siamo prima di tutto interessati, cerchiamo di capire, ma non è detto che ci si riesca. Per esempio, l'emendamento 1.104 propone una sostituzione lessicale: alla «autorizzazione legislativa» propone di sostituire l'«autorizzazione di spesa»; "ed euro" è sostituita con "e di euro". È trasparente fin dall'inizio che la seconda sostituzione riguarda un refuso, ma la prima ci poneva in condizioni di curiosità.

1 le parole «autorizzazione legislativa» con «autorizzazione di spesa». Sono perplesso. Non ho un'opinione precisa, ma sono obbligato a rendere noto all'Aula che si può restare interdetti di fronte a questo tipo di sostituzioni.

temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati».